uscite sulla stampa circa l'incarico che sarebbe stato dato a tale Alessandro Amadori di coordinare un *pool* per la stesura delle linee guida per l'introduzione di una sorta di educazione affettiva ed emotiva nelle scuole per contrastare la violenza di genere. Tale Alessandro Amadori sarebbe autore di un libro in cui si parla di guerra dei sessi, della cattiveria delle donne e della

perché c'è una piccola, ma appariscente popolazione di donne che approfitta della tendenza maschile alla sottomissione per farne una vera e propria fonte di *business*.

provvedimento in discussione reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e del gas naturale, conseguenti alla cessazione, con il terzo trimestre 2023, del meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti disagiati avviato nel quarto trimestre del 2021 e attuato dall'ARERA tramite l'applicazione di compensazioni complementari integrative rispetto al *bonus* base. Il comma 1 prevede che l'ARERA provveda ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre del 2023, in modo tale che per ciascuna tipologia di cliente disagiato i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa siano quelli già previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016 per l'energia elettrica e all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 per il gas, pari al 30 per cento della spesa per l'energia elettrica al lordo di tasse e imposte, e pari al 15 per cento della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte. Il comma 2 dispone che per l'anno 2023 l'ARERA predisponga la relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale entro il 31 maggio 2024. Il comma 3 conferma per il quarto trimestre del 2023 l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Ai relativi oneri, pari a 300 milioni si prevede, a valere sulle risorse già disponibili, presso la cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 4). Il comma 5 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano, in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria. Il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il quarto trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale. Il nuovo contributo opera in luogo di quello precedentemente previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023 a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di *bonus* sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro megawattora. Il vecchio contributo è dunque soppresso e parte delle relative risorse vengono impiegate dal comma 9 per la compensazione dell'onere derivante dal nuovo L'articolo 1-*bis* autorizza i Comuni per la finalità di pianificazione energetica a richiedere all'acquirente unico la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas. L'articolo 2, commi 1 e 3, riconosce un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, i cui oneri sono quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, e prevede che la *social card* possa essere utilizzata, oltre che per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, anche per l'acquisto di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale. Il comma 4 incrementa di 12 milioni di euro per il 2023 il fondo *bonus* trasporti. Il comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro per l'anno 2023, destinati alla corresponsione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022-2023. Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 4 e 5. L'articolo 3 modifica la disciplina delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, alla luce della comunicazione della Commissione europea recante disciplina in materia In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che possano accedere a tali agevolazioni le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a un operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione, individuati come tali dalla citata comunicazione o comunque considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti. È prevista una disciplina transitoria con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo. Restano escluse dall'agevolazione le imprese che, pur in possesso dei requisiti sopra descritti, si trovano in stato di difficoltà (comma 3). I commi da 4 a 7 stabiliscono l'intensità delle agevolazioni riconosciute dalle imprese energivore in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinato al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio. Il comma 8 obbliga le imprese beneficiarie ad effettuare una diagnosi energetica e ad adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il comma 9 affida all'ENEA il compito di effettuare i pertinenti controlli in collaborazione con il GSE e l'ISPRA. I commi 10 e 11 rinviano a successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione delle disposizioni attuative. Il comma 12 attribuisce alla CSEA il compito di trasmettere al MASE, alle Camere e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazione e di provvedere agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato. Si dispone, inoltre, al comma 15, l'incremento della pianta organica della CSEA in cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale. Il comma 13 prevede l'individuazione, da parte del MASE, di un esperto indipendente per la valutazione *ex post* del regime di agevolazioni. Il comma 14 prevede che l'efficacia delle disposizioni in commento sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. L'articolo 4 concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano già state constatate non oltre la data

del decreto legislativo n. 270 del 1999 di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, volta a chiarire che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione

di analisi e valutazione della spesa previste dal decreto legislativo n. 123 del 2011 e non solo, come precedentemente previsto, per quelle relative alle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'articolo 25 del predetto decreto legislativo. Il comma 2 esclude l'applicazione a SIMEST e SACE dei vincoli, dei divieti e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti nei confronti dei soggetti inclusi dall'Istat nel conto economico delle pubbliche amministrazioni. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Restano altresì ferme le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Il comma 3 ammette a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili alcuni interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC,

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

è più di un anno che discutiamo del problema del caro energia, nel senso che ogni tanto si emana un decreto-legge per introdurre o per procrastinare i *bonus* relativi al costo dell'energia.

a quest'Aula che questi lavoratori di certo non si fermeranno: stanno protestando da mesi e stanno vincendo le cause.

oggi tocca a loro perché è la questione più grossa, però questo è un meccanismo che rischia di valere per tutti - e sottolineo

questo provvedimento arriva in un momento particolare dal punto di vista geopolitico, un momento che ha fatto praticamente cadere tutte le ambizioni del piano Mattei. Si diceva che cambiando il fornitore potevamo diventare più indipendenti dal punto di vista energetico e poi ci siamo resi conto che non è così. Non si risolvono i problemi sostituendo il gas della Russia con il gas dell'Algeria

il popolo armeno ha subito un attacco di non poco conto per i civili). Abbiamo visto come i problemi energetici del nostro Paese non si risolvono cambiando lo "spacciatore di caramelle", ma si risolvono andando a cercare tutti gli strumenti che ci consentono di produrre l'energia, che è un fattore chiave per lo sviluppo economico. Oggi senza energia non avremmo questa amplificazione, non avremmo la possibilità di utilizzare i computer e di vedere illuminate le nostre case; non avremmo nulla. Questo fattore così competitivo per lo sviluppo economico del nostro Paese oggi risulta, nei Paesi industrializzati, fra i più cari di tutto il mondo. Noi paghiamo l'energia di più degli altri Paesi e quindi le nostre imprese diventano sempre meno competitive, soprattutto in un periodo come questo che si sta avvicinando a una recessione. Avere quindi un costo di un costo di acquisto dell'energia basso significa anche crescita economica e possibilità di sviluppare le imprese del nostro Paese. questo lo possiamo fare solo puntando sulle fonti rinnovabili, che sono le fonti di energia a più basso costo. Tutti gli studi ormai dimostrano che il costo di queste fonti di energia è sceso molto nel tempo. È logico che parlo dei dati attuali perché trenta anni fa le fonti rinnovabili erano costose. però che ancora molti ragionano con i dati di trenta anni fa. Oggi tutti gli studi rilevano che queste fonti sono disponibili in Italia a basso costo. Tutti gli emendamenti che abbiamo

chiediamo da tempo. Abbiamo visto ad esempio le comunità energetiche. Ogni mese il ministro Pichetto Fratin parla di pochi giorni; vi assicuro che a me lo sta dicendo da quando l'ho conosciuto, dal giorno dell'insediamento di questo Governo.

anno e siamo con oltre un anno di ritardo sulle comunità energetiche. Resto altresì basito quando proponiamo degli emendamenti che non hanno nessun costo. È purtroppo abbastanza demoralizzante

Possiamo tranquillamente chiudere il Parlamento perché tanto non ha alcuna funzione, deve solo ratificare quello che il Governo dice. Sono sicuro che anche voi, senatori della maggioranza, siete mortificati da questo atteggiamento del Governo.

l'emendamento 1.0.5 che chiede soltanto che i distributori comunichino ai Comuni i dati dei consumi dei loro POD POD e dei loro PDR, quindi i dati dei consumi energetici delle scuole, degli uffici comunali e degli asili in maniera elettronica ogni anno. *(Brusìo)*. Presidente, potrebbe chiedere un po' di silenzio perché è difficile parlare?

degli strumenti pianificatori per le comunità energetiche. Oggi i Comuni non hanno nessun dato; spesso devono spulciare centinaia di pagine di bollette per avere qualche indicazione sui consumi energetici *(Applausi)*, quando questi dati sono ampiamente disponibili in Excel dai distributori dell'energia. Abbiamo presentato un emendamento che non costa nulla, chiedendo che questi dati vengano dati ai Comuni, che sono degli enti pubblici, e voi ce lo bocciate. Allora è evidente che non ve li siete letti, è evidente perché un emendamento che non costa nulla, di buon senso che aiuterebbe tutti i Comuni, di centrodestra e di centrosinistra, viene bocciato. Non ha senso continuare a presentare emendamenti che non vengono nemmeno letti da questo Governo. È possibile che su 500 emendamenti non ne vada bene uno? Nemmeno quelli a costo zero? C'è una preclusione nei confronti di questo Parlamento, che cerca di migliorare i provvedimenti che arrivano dal Governo; e questo è inaccettabile. Concludo così; volevo dire altro, ma i miei colleghi mi hanno censurato, perché erano parole troppo forti, e quindi chiudo il mio intervento.

È iscritta a parlare la senatrice Minasi. con il provvedimento oggi in Aula smentiamo, per l'ennesima volta, le critiche strumentali dell'opposizione (ne abbiamo avuto un assaggio ora), che ci accusa di fare solo promesse che non manteniamo e di disinteressarci dei cittadini, soprattutto delle fasce e delle categorie più deboli. Con queste misure infatti, a dispetto delle solite polemiche, ci occupiamo innanzitutto di chi ha più bisogno, alleviando i costi legati al caro bollette, che - come sappiamo - a volte gravano pesantemente, in modo tale da rendere difficile, se non impossibile, arrivare a fine mese per alcune famiglie. Ne discutiamo da oltre un anno, da quando ci siamo insediati, dal momento in cui la guerra in Ucraina ha fatto impennare i prezzi delle materie prime e in particolare quelli per le forniture di energia elettrica e gas. Abbiamo lavorato su più fronti, partendo proprio dal caro bollette e dai rimedi che potessero mitigarlo, aiutando i cittadini non solo e non tanto con piccoli interventi, ma con provvedimenti di largo respiro, sia pure limitati nel tempo; ne seguiranno ovviamente altri, a mano a mano che valuteremo la situazione, così da scegliere di volta in volta quali azioni siano siano migliori e soprattutto in attesa di portare a compimento le misure strutturali su cui il Governo punta per rendere l'Italia autonoma dal punto di vista energetico. Lo sappiamo già, ma è bene ribadirlo anche in questa occasione: il nostro Paese sta scontando scelte miopi di chi, prima di noi, non si è impegnato per investire su politiche che consentissero di superare la dipendenza dell'Italia dall'estero per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, ed anzi, con appositi accordi, ha ancor di più rafforzato tale tale dipendenza, portandoci oggi alla situazione complicatissima che stiamo vivendo a danno dell'intera cittadinanza, che ovviamente ne sconta il prezzo. Dunque, caro senatore Magni, mentre da un lato si agisce sul fronte strutturale, per una nuova politica energetica che porti finalmente a coprire in autonomia il nostro fabbisogno (penso all'idroelettrico, allo sfruttamento delle nostre risorse, ma soprattutto l'insistenza della Lega sul ricorso al nucleare di ultima generazione, che ci fornirebbe energia pulita e sicura a basso costo), parallelamente si interviene con importantissimi sostegni che possono dare fiato non sono alle famiglie, ma anche alle imprese. Prevediamo innanzitutto il rinnovo del *bonus* sociale energia, con l'aggiornamento da parte di ARERA dei valori delle compensazioni applicabili, riuscendo a ridurre le bollette per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro e per le famiglie numerose che abbiano un ISEE superiore a 30.000 euro o familiari in gravi condizioni di salute. Questa misura non credo sia di poco conto. Stanziamo, inoltre, 300 milioni di euro per l'istituzione di un contributo straordinario per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, che cresce in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Prevediamo una riduzione dell'IVA al 5 per cento sul gas fino a fine anno, estendendola anche al teleriscaldamento e all'energia termica, riuscendo così a unificare l'imposta senza disparità di trattamento. Anche per le imprese energivore, adeguiamo le agevolazioni tariffarie alla normativa europea, contrastando la delocalizzazione anche attraverso questa forma, in aggiunta agli altri provvedimenti in materia. Introduciamo, poi, una premialità per le imprese che coprono almeno il 50 per cento del consumo di energia elettrica con quella prodotta da fonti che non emettano carbonio, coniugando così anche rispetto dell'ambiente e l'esigenza della transizione *green*. In questo caso, però, diamo loro il compito di monitorare le emissioni, di adottare ulteriori misure sotto il controllo dell'ENEA e dando mandato al CSEA di trasmettere una relazione al Ministero, alle Camere e all'ARERA sull'andamento del regime delle agevolazioni, così da avere un monitoraggio costante ed evitare anche gli sprechi. Sempre nell'ottica di evitare sprechi e razionalizzare i consumi, come Lega vantiamo un importantissimo emendamento sulla possibilità di pianificare, per i Comuni, le politiche energetiche locali. Questa è una grande novità, che consente innanzitutto di responsabilizzare gli enti locali e, soprattutto, di programmare, nel modo a loro più congeniale, le forniture di energia, secondo una pianificazione ben strutturata, che tenga conto di quali sono le zone e i quartieri più energivori rispetto ad altri. Ma non ci fermiamo qui con le politiche di sostegno ai bisognosi. Destiniamo, infatti, altri 100 milioni di euro ai titolari della *social card* per l'acquisto del carburante e per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto; incrementiamo il fondo del *bonus* trasporti di altri 12 milioni di euro, che si aggiungono ai 110 che già avevamo stanziato in precedenza, come anche il fondo integrativo statale per le borse di studio, di 7,4 milioni di euro, così da aumentare il numero dei meritevoli che potranno accedere alla formazione superiore e che non beneficiano degli aiuti regionali. Prevediamo, poi, la possibilità di un ravvedimento operoso, cui potranno ricorrere i contribuenti che abbiano commesso violazioni nella trasmissione telematica dei corrispettivi nel periodo tra giugno e gennaio 2023, così da aiutare i piccoli commercianti a porre riparo a qualche inosservanza o irregolarità senza andare incontro a guai maggiori avvicinando, quindi, il fisco e lo Stato al cittadino, anziché farlo sempre percepire come un nemico. Infine, anche in tema di spesa pubblica, chiariamo prima di tutto una norma della legge Marzano per il passaggio del complesso aziendale tra Alitalia e ITA, escludendo le due società italiane, coinvolte nelle norme di rilancio della nostra economia *post* pandemia, dai vincoli e dagli obblighi in tema di contenimento della spesa pubblica previsti per i soggetti inclusi dall'Istat nel conto economico delle pubbliche amministrazioni. Soprattutto, ci concentriamo ancora una volta sul PNRR e sul PNC, proprio per garantire la realizzazione degli interventi programmati nei tempi fissati. Diamo, infatti, la possibilità di realizzare alcuni di questi interventi beneficiando del fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti dei costi materiali. In particolare, poi, per gli interventi del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, che hanno aderito ad Accordi Quadro Invitalia, si garantisce una quota aggiuntiva di tale fondo, pari al 10 per cento del contributo assegnato. Quindi, le esigenze primarie del cittadino, quali possono essere sanità e istruzione, vengono anche qui massimamente attenzionate. Vogliamo, infatti, evitare che progetti fondamentali, già stabiliti, finiscano con l'essere cancellati a causa, appunto, dell'innalzamento dei prezzi delle materie prime. quanto descritto non può che convincerci sempre più della bontà del decreto in oggetto, che può dare sollievo alle famiglie, ma anche sorreggere in modo incisivo il sistema produttivo, che sta patendo particolarmente i rincari, che tutti conosciamo purtroppo molto bene, riferibili sia alle sia alle bollette che ai materiali. Pertanto, concludo invitando tutte le forze politiche affinché su tali importanti misure ci siano accordo e unità, soprattutto per il bene dell'Italia e degli italiani.

è l'ennesimo provvedimento *spot* dal titolo ad effetto che il Governo ha blindato con un'ingiustificabile forzatura, confermando la propria avversità al confronto in Parlamento. Nonostante l'importanza degli argomenti trattati, il decreto-legge è giunto in Senato per la conversione in legge senza alcuna possibilità di correggerlo e migliorarlo. Nonostante l'importanza degli argomenti trattati, anche alla Camera il decreto-legge è stato approvato con il voto di fiducia, che ormai è diventato l'arma del Governo per cancellare il dibattito parlamentare e zittire la sua stessa maggioranza, ritenendola politicamente acefala, passiva e supina. Solo per ricordarlo ai colleghi di maggioranza, signora Presidente: scelta oligarchica, errore drammatico, vergogna, mortificazione del Parlamento, deriva democratica e addirittura esproprio delle Camere con cui la presidente Meloni, da deputata dell'opposizione, definiva il ricorso alla fiducia come un assalto alla democrazia. Ci vuole grande sfrontatezza, politicamente parlando, per dimenticare alla svelta quelle posizioni e raggiungere, come avvenuto oggi, il *record* di fiducie poste a danno del Parlamento e degli elettori che lo hanno eletto. L'Esecutivo Meloni si caratterizza per la propria improvvisazione, la propria superficialità e la propria distanza dalla realtà quotidiana di chi vive e opera in Italia. al costo della bolletta elettrica, come Partito Democratico, abbiamo provato a proporre precisi emendamenti per alleviarne il peso per famiglie e imprese, già molto provate dalla crisi. Nel merito, se il Governo avesse accettato il confronto, con questi emendamenti avremmo permesso di sterilizzare gli oneri di sistema e riorganizzarli, in linea con i richiami fatti dall'autorità del settore. Ancora, come Partito Democratico abbiamo proposto il credito d'imposta per le piccole e medie imprese e per gli artigiani, insieme a un fondo di garanzia per realizzare le comunità energetiche rinnovabili, ma anche su questo avete detto no.

ciò che sostiene da un anno, ossia che il Governo sta dialogando con la Commissione europea ed è quasi pronto. La verità è che questi decreti non esistono per incapacità politica, per malafede politica o per entrambi i motivi. Ancora, con un altro emendamento abbiamo proposto la proroga di un anno per il superamento della maggior tutela. L'abbiamo fatto per il grave rischio che nel 2024 le bollette schizzino alle stelle, perché la scadenza del mercato tutelato, fissata al prossimo 10 gennaio, è alle porte. Ciononostante, il Governo è in gravissimo ritardo sulla campagna di comunicazione per informare i cittadini, ha preso tempo, ha eluso il problema e ha vietato il confronto: nel frattempo, la situazione è peggiorata e gli italiani ne pagano le spese. Ancora, con altri emendamenti abbiamo proposto precise agevolazioni per alleviare le difficoltà economiche e sociali nei Comuni già colpiti dalle alluvioni. Anche sulla questione il Governo ha voltato le spalle ai cittadini interessati, confermando la propria miopia politica, la propria insensibilità e la propria indifferenza. Nel merito, l'articolo 1 interviene con aggiustamenti del tutto inefficaci. Il Governo ha previsto bazzecole per categorie di cittadini in difficoltà in ordine al quarto trimestre dell'anno corrente, in sostanza quasi alla fine. Infatti, nel 2024 si annunciano tempi bui sul costo delle bollette. Di conseguenza, il Governo sta aumentando l'ansia e la disperazione dei cittadini, confermando un'irresponsabilità politica senza precedenti. In pratica, l'Esecutivo Meloni sta mettendo una manciata di cerotti su ferite economiche e sociali enormi, rinviando ancora una volta la ricerca di una soluzione strutturale del problema energetico. La verità è che il Governo non ha trovato risorse sufficienti, non le ha cercate e non gli importa di farlo. La verità è che il Governo scarica chi non riesce a sopportare il peso del caro energia. La verità è che il Governo ha rinunciato ad avviare politiche di sostegno reale alle famiglie e ai cittadini. In altri termini, il Governo si è reso sordo e cieco proprio quando l'Antitrust ha multato i colossi dell'energia incolpandoli di aver costretto i consumatori a subire un aumento dei prezzi in contrasto con la protezione normativa già accordata dallo Stato. Inoltre, mentre la crisi economica aumenta, risulta un pannicello caldo la conferma, contenuta proprio in questo decreto, dell'azzeramento per il solo trimestre corrente delle aliquote sugli oneri generali del gas. La stessa valutazione si può fare per la riduzione dell'IVA sul gas metano per usi civili e industriali limitata ai consumi dei soli mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024. Insomma, è il solito tirare a campare del Governo. poi inutili le previste disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, infatti esse non danno né stimoli, né incentivi. Ancora, considerata la prossima probabile impennata del carburante, è veramente misero se non offensivo l'ulteriore contributo ai benefici della *social card* ricavato mediante l'aumento di 100 milioni del fondo per l'anno 2023. La cifra stanziata è bassissima e, peggio ancora, per l'anno venturo non si prevede alcuna speranza. Per inciso, inadeguato e inattuale è l'aumento di quasi 7,5 milioni del del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio legate all'accesso alla formazione superiore. L'aumento poteva e doveva essere maggiore. inoltre soltanto un condono per furbi la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso che il provvedimento in esame ha introdotto per i contribuenti già responsabili di violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi. Insomma, il nostro è un voto contrario contrario e un giudizio contrario per più motivi. Il primo è perché il provvedimento non prevede un aiuto reale ai cittadini; il secondo è per il metodo, che è completamente sbagliato, che offende la dignità dei due rami del Parlamento e rimarca la proverbiale scorrettezza istituzionale del Governo, perché avete impedito l'esame e la discussione del provvedimento e il Governo ha agito da solo, mettendo da parte il Parlamento, calpestandone le prerogative e imponendogli il bavaglio. Il Governo mente su tutto e conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la propria avversione verso l'equilibrio tra i poteri dello Stato e verso il ruolo proprio del Parlamento. diciamo no e votiamo contro per la fiducia che avete posto, perché questo Governo non può meritare la fiducia. Infatti, all'incapacità e all'irresponsabilità dell'Esecutivo si aggiungono la sua intolleranza verso i fondamenti della democrazia e la sua indifferenza nei confronti dei bisogni essenziali dei cittadini. Grazie, consentitemi, in apertura, alcune considerazioni di carattere generale. Quando ascolto infatti alcuni interventi dei rappresentanti del centrosinistra, spesso cerco di capire il motivo di alcune dichiarazioni e di determinati atteggiamenti. Comprendo perfettamente che forze politiche come il Partito Democratico, che hanno governato ben undici anni in queste ultime legislature, spesso senza vincere le elezioni, non avendo ancora metabolizzato la sconfitta, oggi cercano di di deresponsabilizzarsi rispetto alla difficile situazione in cui hanno lasciato l'Italia, cercando di addossare le responsabilità al Governo Meloni. Capisco anche l'irritazione dei rappresentanti del MoVimento 5 Stelle, che nella scorsa legislatura hanno beneficiato di un largo consenso elettorale che si è visto pian piano ridurre a causa dei limiti manifestati nel guidare la Nazione e di mantenere gli impegni presi con gli italiani; ma chi è causa dei propri mali pianga se stesso. Il centrosinistra, nel tentativo di costituirsi una nuova identità, sottovaluta la straordinaria capacità degli italiani di valutare e analizzare la situazione economica e politica che stiamo vivendo e le azioni messe in atto dal Governo in questo primo anno di legislatura. I cittadini hanno perfettamente compreso l'impegno del presidente Meloni e del suo Esecutivo nel superare le difficoltà della Nazione e nel ridare autorevolezza e credibilità all'Italia, soprattutto a livello internazionale. La riprova di ciò è che dopo un anno di attacchi continui al centrodestra, il consenso nei confronti del Governo continua a crescere e questo dimostra come le politiche messe in campo in questo primo anno siano in perfetta sintonia con le necessità degli degli imprenditori, dei lavoratori e dei cittadini italiani. Un aspetto, questo, che viene sottovalutato dal centrosinistra, forse perché chi è abituato a governare senza vincere le elezioni è poco interessato ad ascoltare il pensiero dei cittadini. Non solo gli italiani, ma anche le quattro agenzie di *rating* promuovono l'Italia. Vengono promosse la serietà e l'attenta gestione dei conti pubblici del Governo Meloni, che finalmente riconsegna stabilità alla Nazione, un Governo che mette fine alla politica degli sprechi, quella dei *bonus* a pioggia, dei monopattini, dei banchi a rotelle, per capirci. che, come dimostra la legge di bilancio, concentra le risorse su grandi priorità: sulla crescita economica, sulla sanità, sulla difesa del potere di acquisto delle famiglie, con la conferma del taglio al cuneo fiscale per garantire più soldi in busta paga per i redditi medio-bassi. Il taglio del cuneo fiscale porterà mediamente nella busta paga dei lavoratori circa 100 euro in più al mese che spalmati per tutto l'anno equivalgono a quasi una mensilità in più. Le risorse che si hanno, dunque, sono concentrate su chi ha più bisogno e ne è una riprova il decreto-legge oggi in discussione. Il testo all'esame dell'Assemblea, infatti, è l'ultimo di una serie di provvedimenti che fin dal suo insediamento l'Esecutivo ha dovuto adottare per contrastare le gravissime conseguenze socioeconomiche derivanti dal conflitto bellico in Ucraina, a cui si è recentemente aggiunta la crisi in Medio Oriente. come è sempre accaduto, soprattutto, ci troviamo di fronte a un approccio prudente e realista del Governo Meloni per contrastare il caro energia, un approccio che tiene conto della situazione economica in relazione allo scenario internazionale, ma che allo stesso tempo è sostenibile per la finanza pubblica. Un approccio che concentra gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno delle famiglie, soprattutto quelle più fragili, e a sostegno delle imprese italiane. Il decreto-legge che siamo chiamati ad approvare prevede misure per il contenimento dei costi energetici e interventi per sostenere il potere di acquisto degli italiani, misure per consentire l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale. di conversione si pone due obiettivi principali: da un lato, cerca di risolvere l'emergenza in corso dando risposte rapide in favore dei cittadini e delle attività economiche, dall'altro lato tenta di riportare un equilibrio e una giustizia sociale rispetto a fenomeni economici che si sono manifestati negli ultimi tempi, mantenendo alta la competitività delle imprese italiane e con un occhio di riguardo al merito. Vedremo che tra le misure contenute nel decreto-legge ci sono alcune conferme, come l'implementazione di misure già messe in campo dal Governo Meloni e già operanti in favore dei soggetti più fragili dal punto di vista economico e fisico e a sostegno del loro potere d'acquisto. Si interviene estendendo al quarto trimestre le agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas. Si conferma fino al 31 dicembre l'aliquota IVA al 5 derogando all'aliquota del 10 per cento e del 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente per la somministrazione di gas metano utilizzato per usi civili e industriali. Viene previsto l'utilizzo della *social card* anche per l'acquisto di carburanti o in alternativa di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale mediante un incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione del fondo per l'acquisto di beni di prima necessità destinato alle fasce più fragili dei cittadini. L'attenzione ai più giovani e al merito è resa evidente, invece, con l'incremento di 7,5 milioni del fondo destinato alle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore, per garantire la copertura a tutti gli studenti idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relativo all'anno accademico 2022-2023. Con il decreto-legge, inoltre, vengono disciplinate le agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica. Rispetto a quanto si è detto anche quest'oggi in Commissione, desidero precisare che nel provvedimento non c'è nessun condono. Il ravvedimento operoso concesso ai contribuenti per errori in operazioni avvenute durante la fase dell'inoltro dei corrispettivi elettronici è la semplice dimostrazione di un Governo non ostile al contribuente, che lavora per andare incontro alle attività che generano occupazione ed economia, perché, contrariamente a quanto pensano il centrosinistra centrosinistra e il MoVimento 5 Stelle, la crescita economica non si ottiene per decreto, ma aiutando le imprese, soprattutto quelle in difficoltà. in esame il Governo Meloni conferma la sua vicinanza alle fasce più deboli, agli studenti, alle imprese e alle necessità della Nazione; si interviene con misure adeguate per dare oggi agli italiani quelle risposte che un centrosinistra, sordo all'istanza dei cittadini, non è mai riuscito a dare. Grazie,

Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 937, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131,

Signora Presidente, il ministro Ciriani ha letto la formula di rito e ho deciso che ad ogni fiducia anch'io leggerò una formula di rito: il Parlamento è mortificato e l'opposizione non può dire la sua: una deriva davvero preoccupante per la nostra democrazia. Firmato Giorgia Meloni, 21 settembre

Grazie, Presidente. premetto che ascolto, non accuso e non attacco mai la maggioranza. Quando viene quindi detto che l'opposizione fa queste cose, non mi considero coinvolto e trovo che sia un modo per deviare l'attenzione degli italiani dai veri problemi. trentaquattresima o trentacinquesima questione di fiducia posta dal Governo; praticamente stiamo viaggiando a tre voti di fiducia al mese. Si stanno battendo tutti i *record*. Eppure, a differenza dei suoi predecessori, questo Governo avrebbe dei numeri ampi, ma evidentemente non bastano. Questa costante mortificazione delle funzioni e delle prerogative del Parlamento ha raggiunto livelli intollerabili e contrari allo spirito ispiratore della nostra democrazia parlamentare. Come è intollerabile che un Governo chieda ai propri parlamentari di non presentare emendamenti alla manovra economica, con la conseguenza, quasi divertente, che poi i colleghi della maggioranza quelle proposte le fanno ricadere su altri provvedimenti, oppure vengono da noi delle opposizioni a chiedere la cortesia di farci carico di alcune loro proposte. È chiaro a tutti che questo riflette un problema di ordine politico all'interno della maggioranza, che si registra soprattutto sui provvedimenti economici e fiscali. Lo abbiamo visto la scorsa settimana sulla proroga termini e in quelle ancora precedenti sulla delega fiscale; e lo vedremo - temo - anche nella legge di bilancio. Ad ogni modo, Presidente, noi oggi discutiamo un provvedimento tanto roboante nel titolo, quanto misero nei contenuti. Mancano le risorse, si continua a dire. La verità è che manca la volontà politica di reperirle, attraverso una seria lotta all'evasione fiscale e la messa a terra di politiche economiche che facciano da moltiplicatore economico. Manca un impegno forte per la competitività, che viene sacrificata in nome di un approccio corporativo dettato dai potentati di categoria, dai balneari ai Coldiretti, alle numerose sanatorie, all'introduzione del concordato preventivo con cui si rende legge la iniquità tra i contribuenti. Alla diminuzione del costo dell'energia non è coincisa una diminuzione delle bollette. Il passaggio al mercato libero rischia di tramutarsi in un vero e proprio salasso per le famiglie, anche a causa dei comportamenti sleali e commercialmente aggressivi di alcuni operatori. Cosa sta facendo la maggioranza per evitare che questo accada? Nel frattempo il costo del denaro e quello dei mutui bancari è diventato insostenibile, ma le banche si sono guardate bene dal ridurre le spese sulle giacenze bancarie. Avevate scelto una strada interessante con gli extraprofitti, ma poi avete ingranato una clamorosa retromarcia. E chissà quanti *bonus* sociali e quante bollette si sarebbero potute calmierare con quei tre miliardi. L'inflazione ha duramente colpito il potere d'acquisto delle famiglie e ha ridotto il valore di salari che - è bene ricordarlo - sono tra i più bassi d'Europa. Ma anche qui sono state inscenate ignobili pratiche dilatorie contro il salario minimo, che consentirebbe di affrontare il tema del lavoro povero per tre milioni di italiani. E si potrebbe continuare ancora: che fine ha fatto quel taglio alle accise della benzina che per anni avete venduto come una cosa immediata e fattibile, costruendoci parte delle vostre fortune elettorali? Avete smesso di parlarne, perché nel frattempo le accise sono state rimesse. Non una parola viene spesa a difesa di quelle famiglie che non sono in grado di pagare le rate di prestiti e mutui; a luglio avevano raggiunto complessivi 15 miliardi di euro. Allora, Presidente, noi possiamo parlare di premierato e di legge elettorale, possiamo sciorinare tutto il populismo penale che vogliamo, inventandoci reati a misura di ogni micro-categoria di malefatte. Ma questo non distoglierà gli italiani dalle mancanze di questo Governo e dalla sua incapacità di far fronte ai problemi reali di ogni giorno (il costo della vita, il giro di vite sulle pensioni, il collasso del sistema sanitario), in corrispondenza di un costante calo del potere d'acquisto delle famiglie e di un continuo aumento dei costi per le aziende. Cara maggioranza, se non fate un cambio di passo vero, se il vento non cambia sul serio, ovvero se non metterete in campo una politica economica di sviluppo per la giustizia sociale degna di questo nome, povera Italia e poveri gli italiani, compresi quelli che vi hanno votato. Annuncio pertanto il voto contrario del nostro Gruppo al provvedimento e alla fiducia. Signora Presidente, francamente potremmo incominciare a parlare del fatto che ormai il bicameralismo è soppresso in questo Paese, del fatto che non c'è più un decreto che veda la doppia lettura e conceda al Senato o alla Camera una più completa possibilità di presentare emendamenti, che poi è il ruolo del parlamentare. Potremmo incominciare a dire che questa è l'ennesima fiducia, che forse questo provvedimento non aveva bisogno di fiducia e che così è strozzato completamente il dibattito. Ma voglio incentrarmi sul tema di questo decreto, che viene sontuosamente chiamato decreto energia. Ed io, dunque, mi aspettavo di trovarvi dentro norme che parlassero di energia. Invece, ci sono, sì, delle delle misure che aiutano, in qualche modo, le famiglie a pagare le bollette ed è sempre gradito quando lo Stato cerca di aiutare le famiglie più bisognose a fare ciò. Ma questo provvedimento si esaurisce qui. questo provvedimento si esaurisce qui. Eppure, c'è tanto da fare in tema di energia. Ci sarebbe da rivedere una bozza di decreto che agisca sulle aree idonee. A ogni convegno, i Ministri che intervengono promettono che, da oggi al 2035, verranno autorizzati più di 75 gigawatt di rinnovabili: quest'anno siamo a tre; lo scorso anno erano due. Quindi, come facciamo, da oggi al 2035, a volte tanto? Quando poi abbiamo provvedimenti in bozza che, invece, non consentiranno di fare neanche più un gigawatt, se vengono approvati: diventa antieconomico in alcuni casi, impossibile in altri e, soprattutto, si continua a lasciare uno strapotere alle soprintendenze dello Stato, sia regionali che nazionali, per dire di no in ragione di un bene ambientalmente tutelabile come il paesaggio italiano. Ci sarebbe da aspettare una

prezzi e poi la guerra, successivamente, che il nostro Paese, che è trasformatore, e non produce molte delle materie che utilizza per la propria industria, ha bisogno di avere una certezza certezza energetica. Invece questa certezza non c'è e non ce la daranno gli accordi che abbiamo fatto con altri Paesi che, per carità, hanno sostituito temporaneamente la Russia, ma che non hanno quella stabilità politica e quella democrazia che ci permette di dire che abbiamo svoltato e abbiamo dato sicurezza alle nostre imprese. Mi aspettavo, banalmente, una strategia su un'energia come

ormai da troppo tempo. Io mi auguro, veramente, che sia il ministro Pichetto Frattin sia il ministro Urso dicano dicano che cosa vogliono fare per il nostro Paese in tema energetico e lo dicano prima di tutto agli imprenditori che si occupano di energie alternative; imprenditori che hanno bisogno di certezze e troppe volte lamentano che continuamente cambiate le norme, le misure che loro devono attuare, e non riescono a fare una programmazione pluriennale. Questo, per un'impresa, è qualcosa di drammaticamente pesante. Vorremmo sapere, banalmente, quando arriverà il provvedimento sulle comunità energetiche: Se ne fa un gran parlare, sempre appunto nei convegni, e poi non si possono realizzare; quando e come si realizzeranno tutte le misure promesse nel PNRR o se pensate di far ritornare indietro le risorse anche su questo capitolo. Insomma, avremmo voluto sentire parlare di energia. Per motivi che noi ignoriamo - ogni volta viene promesso un decreto energia-*bis*, sui giornali o nelle conferenze stampa - in Consiglio dei ministri questo decreto non arriva mai. Vorremmo sapere, banalmente, se per l'idroelettrico e le concessioni ci sarà una proroga; se ci sarà una proroga affinché le famiglie, anche quelle non fragili, non entrino nel mercato non tutelato. Insomma, sono molte le domande che avremmo voluto fare e forse avremmo avuto anche alcuni emendamenti da proporre. Avverto che in Commissione non ho neanche tentato di fare quello che in maniera giusta i miei colleghi hanno fatto, presentare emendamenti, perché mi sembrava una presa in giro doverli fare nel giro di un'ora e in altrettanto tempo vederli praticamente bocciati. Pertanto, dichiaro il voto contrario a questo ennesimo voto di fiducia, lanciandovi una sfida: quando vorrete parlare di energia, ci saremo, con le nostre competenze e le nostre idee, sperando che ci vogliate ascoltare e non vogliate strozzare ancora una volta il dibattito in pochi minuti, tra una fiducia e l'altra, in una Camera sola. Così non si fa bene al Paese e rimangono inevase molte delle sollecitazioni che gli *stakeholder* pongono a noi e immagino vorrebbero porre a voi, con emendamenti puntuali. Per questo il nostro voto è contrario e speriamo che la prossima volta vada meglio. *(Applausi)*.

dell'ennesimo decreto-legge che segue una prassi democraticamente scorretta e pericolosa per il Paese, tanto che nuovamente la maggioranza è qui a chiederne la votazione a scatola chiusa. È questa la modalità operativa che ci troviamo ad affrontare anche oggi, del tutto finta e soprattutto ipocrita nei confronti di cittadine e cittadini, da cui noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra ci dissociamo completamente. Anche questa volta mancano del tutto le garanzie che permettano un'approfondita analisi e un sano confronto su questo decreto-legge relativo al caro prezzi dell'energia. Mancano i passaggi fondamentali in Commissione, manca di nuovo il relatore in Aula. Ormai non si prova nemmeno più imbarazzo a chiedere ai Gruppi parlamentari di presentare gli emendamenti entro un'ora dall'incardinamento del disegno di legge in Commissione. Questa strategia e questo *modus operandi* rappresentano un vero e proprio insulto all'Italia democratica, al nostro lavoro e anche a quello svolto dai nostri nostri eccellenti uffici legislativi. Così, anche oggi dobbiamo assistere alla solita pantomima, ormai nemmeno più ben recitata, che consuma e riduce il potere emendativo e deliberativo di questo Parlamento a pura farsa; metodo che la maggioranza di Governo non ha problemi a seguire, ma a cui io personalmente non mi abituerò mai. Questo decreto calderone, che oggi ci state chiedendo di convertire in legge, proprio per la fretta con cui deve passare - una fretta spacciata per oculato dinamismo, ma che in realtà si rivela di nuovo pessima consigliera - raccoglie norme confuse, senza capo né coda, con le quali pretendete di risolvere le emergenze strutturali di questo Paese. un approccio frettoloso e impreciso, che si snoda attraverso una sequela disordinata di *bonus*, quasi fossero tessere a punti premio da distribuire, fino al loro esaurimento, con in fondo l'eco di ricchi premi e *cotillon*: tutti incentivi provvisori e insufficienti che non riescono a soddisfare nemmeno il fabbisogno primario urgente delle fasce più deboli della società, a cui giustamente sono indirizzati; cerotti temporanei e inefficaci che, anziché puntare a risolvere il problema, lo aggravano nel tempo e da tempo. È il caso del vostro decantato *bonus* sociale elettrico, strumento che per faciloneria avete scelto rispetto alla possibilità da noi richiesta di stabilizzare il prezzo dell'energia sul mercato e con il quale elargite un ulteriore contributo straordinario per i destinatari a copertura degli ultimi tre mesi dell'anno. O forse dovremmo dire delle ultime tre settimane, dato che siamo a fine novembre? Stessa cosa per il *bonus* trasporti, per il quale nel testo oggi posto in votazione prevedete ulteriori 12 milioni di euro nel 2023, che sta terminando, da sommarsi ai 100 milioni previsti per lo stesso anno, cifra comunque sempre inferiore di circa 68 milioni rispetto a quella stanziata dal Governo Draghi. Il fondo istituito è di per sé già ridicolo, se pensiamo a quanti milioni di cittadini, inclusi bambini e ragazzi, usufruiscono quotidianamente del trasporto pubblico in Italia, ma non solo. A beneficiare di questo esiguo *bonus* di 60 euro quale spesa massima *pro capite* finanziata per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto pubblico saranno solo le cittadine e i cittadini con un reddito complessivo non superiore ai 20.000 euro. Anche il limite di reddito è già stato drasticamente abbassato l'anno scorso rispetto alla soglia precedente, che era invece di 35.000 euro. A questo punto anche quest'anno chiedo al Governo se conosca i costi effettivi degli abbonamenti ai mezzi pubblici delle nostre città, utilizzati da tante famiglie per mandare a scuola i propri figli. Questo sempre a copertura solo delle prossime settimane che ci separano dal 2024. Nella tempesta che ci stiamo trovando ad affrontare, tra crisi climatica, terribili guerre e catastrofi umanitarie, continuate irresponsabilmente a navigare a vista e pure a occhi chiusi, senza porvi il minimo problema di come affrontare in modo coraggioso e strutturale il terribile contesto politico e climatico che stiamo vivendo. misure puntuali fini a se stesse, completamente prive di una visione di lungo periodo, sintomatiche di un atteggiamento di totale chiusura rispetto alla necessità di favorire la transizione energetica. Anche in questo provvedimento non c'è traccia di misure per promuovere la sicurezza energetica e la riforma del mercato elettrico, tassello fondamentale per favorire nuove tecnologie di energia rinnovabile. Contro ogni logica e contro ogni buon senso si introducono agevolazioni per le imprese fossili a forte consumo energetico, finanziate con gli incentivi previsti per le fonti di energia rinnovabile: oltre al danno, la beffa. Poco incisivo è infatti il dispositivo-contentino con cui subordinate l'accesso a tale agevolazione per le aziende che riducono l'impronta di carbonio solo per il 30 per cento del proprio fabbisogno energetico e che spendono almeno il 50 per cento di risorse in progetti che abbattono le emissioni di gas a effetto serra. Vi abbiamo proposto delle percentuali più ambiziose, che ovviamente sono rimaste nel cassetto. Si tratta di scelte obsolete e incoerenti rispetto agli impulsi all'innovazione di cui ha bisogno questo Paese e che identificano la visione a corto raggio di questa maggioranza che si rifugia nella politica fittizia dei *bonus* e non in quella proattiva della crescita ambientalmente ed energeticamente sostenibile. Nel settore energetico questa prerogativa di crescita sostenibile e di spirito innovativo in Italia stanno dimostrando di averla soltanto gli imprenditori e le realtà industriali lungimiranti, e direi per fortuna: fuori c'è un'Italia molto più avanti della classe politica che sta governando il Paese. Senza scomodare Mattei, tante e diverse imprese virtuose italiane sono passate eccellentemente dal paradigma fossile a quello delle fonti di energia rinnovabile, ottimizzando i tanti consistenti benefici economici di una transizione energetica che va oltre qualsiasi ideologismo. Purtroppo non solo questa prerogativa continua a essere assente tra i decisori politici, ma non si manifesta neppure la consapevolezza di quanto potrebbe essere decisiva la scelta di intraprendere seriamente la strategia della trasformazione sostenibile in tutti i settori dell'economia. Anzi, proprio in quest'Aula si sostiene addirittura il contrario, manifestando senza nessun ritegno la classica noiosa litania dell'ideologismo ambientalista, che francamente ha scocciato. Bisogna definire rapidamente e seriamente come affrontare la gestione ottimale del programma energetico italiano. Inoltre, come da costume di questa maggioranza, sia l'articolo 4 che l'articolo 6 di questo provvedimento introducono delle norme del tutto estranee al tema del caro energia di cui dovrebbe Infatti, l'articolo 4 prevede che coloro che, dal 1° gennaio 2022 al 30 gennaio 2023, non hanno emesso scontrini fiscali o documenti di trasporto o coloro che hanno trasmesso fatture con dati incompleti o non veritieri possono comunque avvalersi del ravvedimento operoso e mettersi in regola attraverso il pagamento di una sanzione ridotta. Qui, oltre ad avere i *bonus*, siamo di fronte a una vera e propria sanatoria nei confronti di chi non ha rispettato gli obblighi dichiarativi dei guadagni ottenuti. una misura che premia ingiustamente coloro che non rispettano la legge, rispetto ai professionisti che dichiarano in modo trasparente ogni minimo guadagno. Anche questa maggioranza continua la saga tutta italiana di premiare i furbi e di penalizzare i fessi - come direbbe Totò - ossia gli onesti. Pure da questa inaccettabile azione noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra ci dissociamo nettamente. Anche l'articolo 6 reca una disposizione che nulla ha a che fare con il caro energia in quanto disciplina l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo in tal senso una disposizione che danneggia i lavoratori e le lavoratrici che vi sono impiegati. Da oggi la cessione di complessi aziendali o dei complessi di beni e contratti prevista da programmi di liquidazione delle imprese in crisi non garantirà il mantenimento dei contratti di lavoro e dunque il trasferimento di coloro che vi lavoravano precedentemente. Una norma lesiva dei diritti dei lavoratori e favorevole alle operazioni di mercato delle grandi società che così facendo non avranno l'obbligo di garantire le giuste tutele ai lavoratori delle aziende in crisi che acquistano, lavoratori che da oggi in poi si troveranno dunque senza impiego e salario. Poi il Governo reagisce stupito e meravigliato se vengono indetti giusti scioperi di lavoratrici e lavoratori, inveendo come da copione contro i sindacati, noncurante del fatto che i problemi hanno radice proprio nelle politiche del Governo che sta bloccando di fatto lo sviluppo sostenibile del Paese. Da ultimo, esule dai temi di questo decreto, ma importante da sottolineare per far comprendere in che direzione si muove la pericolosa politica pseudo-ambientalista di questo Governo, è la costituzione di una commissione interministeriale incaricata di riscrivere la normativa in materia ambientale. Peccato che il Governo voglia nominare soggetti esponenti delle *lobbies* del petrolio e del cemento a far parte di questa commissione, soggetti che dovranno occuparsi da vicino di norme in materia di inquinamento, tutela paesaggistica e di transizione energetica, temi delicati dagli interessi economici miliardari. Questo apre degli scenari preoccupanti sul futuro che ci attende in materia ambientale. Chiediamo al Governo di abbandonare la retorica della propaganda e di assumere un comportamento responsabile e coraggioso per far crescere in maniera sostenibile il nostro Paese. Urge un vero cambio di rotta per il Paese e per le future generazioni. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, forti delle nostre proposte, bocciate senza essere mai state prese seriamente in considerazione, esprimiamo voto contrario su questo provvedimento regressivo.

sul tema dell'energia abbiamo gli occhi ben aperti, non gli occhi chiusi. Li abbiamo talmente ben aperti su questo tema che il testo che è oggi in esame è in assoluta continuità con quanto fatto sinora dal Governo a sostegno delle famiglie e delle imprese per affrontare la crisi energetica e il conseguente rincaro delle bollette ed è stato oggetto di un lungo lavoro parlamentare da parte della Camera dei deputati, che lo ha esaminato e integrato. Il sostegno Il sostegno al potere di acquisto e al reddito netto delle famiglie è stato un punto fermo dell'azione di questo Governo, che sta trasformando in fatti quanto era previsto dal programma elettorale del centrodestra. Sapevamo che gli oneri derivanti dal conflitto russo-ucraino sarebbero continuati in un mercato dell'energia che è stato colpito anche in larga parte dalle speculazioni. Le ulteriori instabilità politiche in Medio Oriente sul fronte del conflitto Israele-Gaza ha creato ulteriore incertezza sui mercati delle *commodities*. L'Italia ha già intrapreso un percorso di riconversione delle fonti energetiche e un'accelerazione verso le fonti rinnovabili, con l'obiettivo dell'indipendenza energetica, ma non possiamo trascurare quanto esiste oggi e nemmeno le conseguenze che ha avuto un'organizzazione delle fonti energetiche basata largamente sul gas di importazione dalla Russia.

un decreto aiuti. I principali destinatari delle misure sono le famiglie e in particolare quelle più bisognose, cioè quelle con i figli a carico o con soggetti disabili che fanno parte del nucleo familiare. Il *focus* di questo decreto-legge è principalmente quello di tutelare il potere di acquisto delle famiglie e quindi dare continuità ai sostegni e agli aiuti che sinora erano stati previsti. Vengono quindi confermati attraverso ARERA i cosiddetti *bonus* sociali, per fare in modo che soprattutto per gli utenti più bisognosi venga mantenuta la riduzione della spesa prevista. Anche per il quarto trimestre di quest'anno continua a essere previsto l'annullamento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas, così come viene confermato per clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, che cresce con il numero di componenti del nucleo familiare, secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale. È stata rifinanziataanche la cosiddetta *social card*, che consente ai titolari l'acquisto di carburante, oppure, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto, così come viene rifinanziato anche il fondo *bonus* trasporti. Vi sono poi altre misure diverse, sempre di carattere sociale: tra queste il rifinanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore, la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per le somministrazioni di gas interno. È poi previsto l'istituto del ravvedimento operoso, con dei limiti temporali precisi per quei contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi. Vengono poi previste procedure per consentire di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi del materiale da costruzione, quindi alcuni interventi del PNRR e del PNC possono essere rimessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Sono previste agevolazioni tariffarie anche a favore delle imprese cosiddette energivore, cui accedono quelle che hanno un consumo di energia elettrica non inferiore a un gigawatt che operino in settori ad alto rischio di rilocalizzazione, oppure che possono essere considerate tali in base a determinati parametri. Insomma, le agevolazioni riconosciute alle imprese energivore in forma di esenzione parziale dal pagamento delle componenti degli oneri generali afferenti al sistema elettrico vengono destinate al sostegno delle fonti rinnovabili. Si introduce anche una premialità per le imprese che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con l'energia prodotta da fonti che non emettono carbonio. Queste devono inoltre adottare ulteriori misure volte a ridurre le proprie emissioni di *green house gas*. Insomma, si tratta di un insieme di agevolazioni rivolte sia ai cittadini, specie quelli più bisognosi, che alle imprese che sono stati più colpiti da questa ondata di rincari energetici. un decreto-legge a cui ha lavorato in gran parte il nostro ministro Pichetto Fratin insieme agli altri ministri del Governo che hanno firmato il testo. Si tratta di norme che assolutamente devono essere convertite in legge ed è per questo che i senatori di Forza Italia voteranno convintamente a favore della fiducia al Governo, soprattutto per questo percorso coerente e lineare a sostegno delle nostre famiglie e delle nostre imprese.

Signora Presidente,io mi auguro che ai colleghi della Lega non dispiaccia il colore del completo che indosso oggi, perché dirò cose scomode, ma ho scelto un colore diverso dal nero e l'ho fatto appositamente per non impressionarli. In apertura di questo mio intervento mi preme innanzitutto sottolineare l'ottimo lavoro svolto dalla maggioranza di Governo nella scelta dei titoli da dare ai provvedimenti, perché a leggere i titoli di quello che approvate in Consiglio dei ministri date davvero l'impressione di occuparvi dei problemi dei cittadini. Il problema è che, presi forse dalla fase di euforia del titolo azzeccato, lasciate questi provvedimenti sostanzialmente vuoti nei contenuti, oppure in contrasto con gli *spot* ai quali ci avete di fatto abituati. Tuttavia degli *spot* e della vostra concezione di merito dirò in seguito, perché sono argomenti che è giusto approfondire in questa sede. Andando al contenuto di questo ennesimo decreto-legge, che avete chiamato misure contro il caro prezzi energia in aiuto a famiglie e imprese, balza immediatamente agli occhi, anche ai meno attenti, come lo stesso provvedimento sia privo di azioni concrete e si allontani in maniera evidente dagli scopi che si prefigge uno dei tanti giochi di prestigio a cui ci avete abituati. Alla Camera avete assicurato il non ricorso alla fiducia, ma poi ci avete ripensato; al Senato avete ben pensato di anticipare l'arrivo del decreto stesso con la volontà di porre la fiducia. Quello che mi chiedo e vi chiedo di spiegarmi è perché diavolo vi vantate così tanto di avere la prima maggioranza votata e voluta dal popolo, una maggioranza assai consistente, e continuate ad evitare il confronto con le opposizioni. Ad essere maliziosi, colleghi, si potrebbe pensare che sia una mossa volta a tenere buoni voi stessi, piuttosto che noi delle opposizioni. *(Applausi)*. La mia ovviamente è una domanda retorica. Sappiamo bene quale sia la vostra idea di democrazia parlamentare: l'avete messa nero su bianco su un disegno di legge che presto discuteremo qui in Senato. Abbiate almeno il coraggio di enunciare quello che è l'assioma della vostra maggioranza: il Parlamento vi piace se dice e fa quello che voi pensate e desiderate. Il testo che votiamo oggi è per certi versi sorprendente. Lo è per quello che c'è, ma anche e soprattutto per quello che non c'è al suo interno e lo è nella misura in cui siete riusciti ad inserire in un provvedimento emanato con lo scopo di andare incontro alle difficoltà di famiglie e imprese alcune chicche e alcune perle frutto della vostra proverbiale concretezza e capacità di andare incontro alle istanze di cittadini e sistema produttivo. produttivo. Partiamo da quello che non c'è: la proroga del mercato tutelato. Bravissimi, la gente non vedeva l'ora di pagare qualcosa in più in bolletta. Decidete di lasciare per strada 10 milioni - e dico 10 milioni - tra famiglie (comprese quelle definite vulnerabili) e imprese, che dovranno passare al mercato libero dopo che voi li avete illusi con la promessa di una proroga, proprio in questo decreto, che non c'è. Con l'articolo 6 date uno schiaffo ai lavoratori Alitalia, provando a bloccare per vie traverse i ricorsi in tribunale per il mancato trasferimento a ITA. Fate una cosa che non ha precedenti nel nostro ordinamento; come vi abbiamo già segnalato in Commissione, la norma da voi messa in campo si configura come un vero e proprio abuso giuridico, perché norma interpretativa, e ciò al solo fine di godere di quella efficacia retroattiva che solo eccezionalmente può concedersi ad una norma giuridica. Con i numerosi *bonus* spostate le risorse senza approntare misure concrete di contrasto al caro energia, senza contare che l'arco temporale delle misure contenute nel decreto è particolarmente breve. Quindi, non avete una strategia energetica, non avete lo sguardo al futuro e, anzi, lo rivolgete esclusivamente alle prossime elezioni, perché siete perennemente in campagna elettorale *(Applausi)*. Con voi nessuna politica energetica, nessun piano per la transizione energetica; anzi, mettete l'accento ancora una volta sul fossile. Signora Presidente, mi faccia far riferimento a ciò che ho ascoltato negli interventi prima del mio. Non accettiamo i riferimenti fatti da una collega della maggioranza: non accettiamo la lezione che i colleghi della maggioranza ci vogliono dare, quando dicono che i Governi precedenti a questo non hanno fatto abbastanza per la diversificazione dell'approvvigionamento energetico. Ricordatevi per quale motivo e per quale volontà le comunità energetiche sono normate e diteci chi è che sta perdendo tempo nell'emanazione dei decreti attuativi. è? Chi ha provveduto all'efficientamento energetico delle abitazioni? Chi è stato a fare questo e chi, ancora, è stato a bloccare questa operazione? Questo mi premeva dirlo, Presidente. Poi c'è l'articolo 4, che avreste dovuto mettere alla fine del testo, perché è un po' la vostra firma. Aiutiamo il Paese in difficoltà con un bel condono per chi non ha rispettato le regole. Anche qui è bello il titolo: «Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi» che, a leggerlo, non fa una piega, anzi. Per chiarezza e correttezza avreste dovuto però rubricarlo come agevolazioni e aiutini per i furbetti del cartellino, che sostanzialmente generano la classica definizione di cittadini di serie A e cittadini di serie B. Si tratta infatti di un condono. È però tutto normale, siete pur sempre voi e non ci stupite più. Signori della maggioranza, ci avete sempre additati come quelli scappati di casa, impreparati e incompetenti. Per voi siamo stati e siamo tuttora un'anomalia; è questa una cosa di cui siamo fieri proprio perché traccia un solco invalicabile tra il vostro e il nostro modo di intendere il servizio al Paese. Vi abbiamo fatto e vi facciamo paura e ne conosciamo bene le ragioni; siamo entrati nei Palazzi, anche in questo Palazzo, senza cognomi altisonanti e voi vi siete persi, vi siete smarriti. Per voi noi siamo senza cognome - lo ripeto - e a voi questa cosa dà fastidio perché avete difficoltà a riconoscerci, perché il sistema di cui voi fate fieramente non ci riconosce e ci vede come un corpo estraneo. È proprio sui cognomi che ultimamente avete fatto un'operazione meravigliosa, degna della peggiore prima Repubblica, ma senza l'abilità di far passare sotto traccia le manovre fatte; abilità che invece concretizzava quella classe politica.

Siete scivolati sui cognomi. Ricordiamo tutti il bellissimo discorso *spot* della presidente Meloni sul merito. Diceva la Presidente del Consiglio la competenza e il merito sono due valori aggiunti per la nostra Nazione. Continuava dicendo: «Noi abbiamo scelto di lavorare per riattivare l'unico ascensore sociale di cui davvero disponiamo, che Affermazioni che, lì per lì, hanno suscitato un plauso, salvo poi renderci tutti conto immediatamente, sin da subito, di aver frainteso quelle parole. La presidente Meloni ha parlato dell'importanza del merito, ma in tutta evidenza si riferiva a quel noto prodotto usato per inamidare le camicie da consiglio di amministrazione, amministrazione, da chiamata diretta, da incarico ottenuto di sorelle, cognati, fratelli, figli, nipoti e parenti tutti. Alla faccia dell'ascensore sociale, che vi piace tanto citare dall'attico della vostra arroganza e della vostra ipocrisia. Altro che norme sulle bollette e in aiuto a famiglie e imprese. Voi state togliendo energia al Paese e lo fate anche dilapidando i soldi ottenuti da Giuseppe Conte in Europa, un patrimonio e un'occasione mai avuti prima. *(Applausi)*. Dovreste vergognarvi e prima o poi - dico prima o poi - dovreste renderne conto se non alle vostre coscienze, almeno al popolo italiano e a quanti hanno creduto alle vostre spudorate spudorate menzogne. Signora Presidente, per questi motivi annuncio il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle a questo ennesimo provvedimento farsa.

Grazie, Presidente. È un provvedimento fondamentale per sostenere famiglie imprese italiane per fronteggiare le gravissime conseguenze

per fronteggiare le gravissime conseguenze socio economiche derivanti dal conflitto bellico in Ucraina, a cui si è aggiunto quello del Medio Oriente, in un contesto già parecchio provato dalla pandemia. La storica politica energetica del nostro Paese ci vede molto svantaggiati rispetto ai Paesi europei, soprattutto a quelli confinanti che beneficiano di prezzi dell'energia molto inferiori non solo grazie al nucleare, ma grazie anche ad accordi commerciali che gli permettono di vendere a noi l'energia elettrica prodotta. È necessario quindi un cambio di rotta che porti il Paese verso una maggiore autonomia energetica attraverso lo sfruttamento delle nostre risorse naturali e investendo su fonti energetiche sicure, innovative e all'avanguardia. Nel frattempo però dobbiamo aiutare imprese e famiglie con provvedimenti di urgenza mirati, come questo che ci accingiamo ad approvare. Non è una norma isolata, bensì un decreto-legge che serve per affrontare un'emergenza relativa all'ultimo trimestre 2023. Ovviamente poi ci saranno altri provvedimenti come questo, altrettanto concreti e coraggiosi. Questa norma introduce elementi importanti: un incremento di 12 milioni di euro sul fondo del *bonus* trasporti, che si aggiunge ai 100 milioni già stanziati. Una misura rivolta alle famiglie, agli studenti e ai lavoratori a basso reddito, che prevede un contributo fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto locale, regionale, interregionale e nazionale. Il provvedimento rifinanzia con ulteriori 100 milioni di euro per il 2023 la carta "Dedicata a te", per i nuclei familiari con almeno tre componenti e ISEE fino a 15.000 euro, che potrà essere utilizzata anche per l'acquisto di carburante. Si incrementa infine di 7 milioni e mezzo di euro il fondo per la concessione di borse di studio per il 2023, destinato a sostenere l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari delle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022-2023. Viene riconfermata la riduzione dell'IVA per le somministrazioni di gas metano per usi sia civili, sia industriali. È stato prorogato l'azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l'aliquota IVA ridotta al 5 per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas metano. Importante è anche l'approvazione dell'emendamento che prevede la possibilità di pianificazione a livello territoriale e comunale (quindi a livello degli di quelle che devono essere le politiche energetiche locali; in questo modo è possibile per i Comuni informarsi su quali siano le zone e i quartieri più energivori rispetto ad altri e di conseguenza sviluppare la pianificazione di merito. Vengono introdotte misure per il contenimento della spesa per le società pubbliche, prevedendo l'esclusione di SIMEST e SACE, che sono le società italiane coinvolte nelle norme di rilancio della nostra economia fin dal momento post-pandemico, dai vincoli e dagli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica. Viene data inoltre la possibilità di realizzare gli investimenti del PNRR e del Piano nazionale complementare utilizzando il fondo per l'avvio delle opere indifferibili, per fronteggiare l'aumento di costo dei materiali, senza dover cancellare progetti già vagliati. Presidente, concludo. I nostri provvedimenti nascono da una politica di ascolto e dal contatto con il territorio e, a differenza delle opposizioni, che fanno giustamente il loro mestiere, dicendo che tutto ciò che facciamo noi non va bene e andando in piazza a protestare contro il Governo (ne risponderanno poi agli elettori), noi lavoriamo per tutelare le famiglie, con un aiuto per pagare le bollette e per arrivare a fine mese. O a differenza dei sindacati, alcuni (i soliti) e fortunatamente non tutti, che hanno provato a bloccare il Paese, ma, grazie all'impegno del ministro Salvini, non ci sono riusciti,

È un paradosso, perché questo è un Governo politico che può contare su un'ampia maggioranza politica, sia alla Camera che al Senato. Ma tutto questo evidentemente non basta e ci tocca assistere anche oggi al voto di fiducia su un decreto assolutamente eterogeneo nei suoi contenuti, che ha seguito un *iter* di monocameralismo alternato, che è ormai diventato la prassi del nostro modo di legiferare. Si va avanti a decreti-legge, li esamina realmente solo un ramo del Parlamento (in questo caso la Camera dei deputati) all'altro ramo è riservato una esame frettoloso (poche ore) e una ratifica senza l'approvazione di alcun emendamento, nella maggior parte dei casi con il ricorso al voto di fiducia. Me lo lasci dire, signora Presidente: non possiamo andare avanti così. *(Applausi)*. Non possiamo andare avanti comprimendo e umiliando il ruolo del Parlamento, come sta avvenendo a colpi di decreti in questa legislatura. E lo dico in una fase in cui la maggioranza ha iniziato a parlare di riforme costituzionali, di premierato, di un diverso equilibrio tra Governo e Parlamento. Gli equilibri tra Governo e Parlamento sono già saltati e se mai si dovesse fare una riforma costituzionale, bisognerebbe ripristinare il ruolo centrale del Parlamento, un ruolo reale, di indirizzo, di controllo, di legiferazione che da tempo, purtroppo, il Parlamento ha parzialmente perso. Veniamo al merito di questo decreto-legge. Il titolo del provvedimento al nostro esame è ambizioso: misure urgenti in materia di energia e interventi per sostenere il potere d'acquisto e tutela del risparmio. In effetti, signora Presidente, il tema del potere d'acquisto è realmente importante. Negli ultimi due anni l'indice dei prezzi al consumo nel nostro Paese è cresciuto di quasi il 15 per cento. Sono tassi di aumento dei prezzi che non vedevamo dalla metà degli anni Ottanta. Nello stesso periodo, le retribuzioni lorde sono cresciute di meno del 6

l'aumento dei prezzi è stato superiore per le famiglie in condizione socio economica maggiormente disagiata. Che cosa ha fatto, signora Presidente, il Governo Meloni di fronte a questa situazione difficilissima, che ha messo milioni di famiglie nella condizione di dover scegliere se pagare le bollette o fare la spesa? Il Governo, con uno dei suoi primi atti, ha eliminato il taglio delle accise deciso dal Governo Draghi per contenere i prezzi del carburante e ha varato un decreto, pomposamente denominato decreto trasparenza, che prevedeva una serie di misure che sono rimaste sulla carta. prevedeva la riduzione automatica delle accise sui carburanti in caso di crescita dei prezzi al di sopra di un determinato livello:

signora Presidente. Quel decreto trasparenza prevedeva i doppi cartelli come misura straordinariamente efficace, nelle intenzioni del Governo, per contenere i prezzi dei carburanti: doppi cartelli che sono stati bocciati, sospesi nella loro applicazione dal TAR del Lazio, con una sentenza di pochi giorni fa, Questa è la triste fine di quel decreto trasparenza. Il Governo ha varato pomposamente quello che ha chiamato il "carrello tricolore", sei mesi dopo un analogo accordo fatto dal Governo francese, quando i buoi erano scappati dalla stalla. *(Applausi)*. Oggi Altroconsumo ci informa che quasi tutti i prodotti oggetto del carrello tricolore erano già in promozione. livello dei carri armati di Mussolini. Si spaccia per carrello tricolore la promozione di beni e servizi che erano già in promozione nella grande distribuzione. Che cos'è questa, se non una presa in giro dei consumatori italiani? *(Applausi)*. Ora arriva questo decreto, recante misure per sostenere il potere d'acquisto. Che cosa prevede questo decreto? decreto? La proroga di alcune misure che erano già state varate a suo tempo dal Governo Draghi: gli oneri di sistema per il gas, l'IVA sul metano, il teleriscaldamento e, all'articolo 2, quella che si configura come una vera e propria presa in giro degli automobilisti italiani. Essi hanno dovuto sopportare un maggior carico di miliardi di euro per effetto dell'aumento dei prezzi dei carburanti nei mesi estivi, con miliardi di euro incassati dal Governo sotto forma di maggiori accise IVA. Le stime parlano di cifre superiori a due miliardi di euro. E quanti di questi soldi il Governo restituisce? Udite, udite: 100 milioni di euro caricati sulla carta sociale *(Applausi)*, un'elemosina caricata su un'altra elemosina, e 12 milioni di euro di rifinanziamento del *bonus* trasporto pubblico, che - ricordiamolo - era stato introdotto dal Governo Draghi su proposta del ministro Orlando, con 190 milioni di finanziamento e una soglia ISEE di 35.000 euro; il Governo Meloni, appena arrivato, ha ridotto il finanziamento a 100 milioni e ha abbassato la soglia ISEE da 35 a 20.000 euro. Vi siete accorti - tardi - che comunque il *bonus* per l'abbonamento al trasporto pubblico era molto richiesto dagli italiani, nonostante l'abbassamento della soglia ISEE, e adesso ci mettete un *cip* di 12 milioni di euro che comunque non basterà: non basterà a dare un'alternativa alle persone che si devono spostare per lavorare e per studiare; non basterà a effettuare quell'investimento sul trasporto pubblico locale che il Governo avrebbe il dovere di fare, nel momento in cui molti milioni di italiani pagano il carburante a prezzi molto più elevati e fanno molta più fatica a spostarsi per lavoro e per studio. Ci sono poi due misure che sono grandi assenti in questo decreto-legge pomposamente chiamato decreto per il potere d'acquisto: le norme attuative per le comunità energetiche, le grandi dimenticate, che sarebbero una straordinaria opportunità per questo Paese, ma che sono nel dimenticatoio, mentre l'Italia potrebbe in poco tempo utilizzare al meglio la prospettiva di una misura che in Germania ha consentito l'attivazione di migliaia di esperienze del genere. E manca soprattutto, signor Presidente, la proroga del regime di maggior tutela per luce e gas, che non è una tecnicalità *(Applausi)*, ma riguarda 10 milioni di famiglie di questo Paese che, se le cose non cambiano, come continuiamo a chiedere, se non viene prorogato il regime di maggior tutela, passeranno al libero mercato - passaggio non preparato a dovere dal Governo - dall'inizio del 2024. Sapete a che livello sono oggi i prezzi medi dell'elettricità sul mercato libero? Sono del 30 per cento più elevati rispetto a quelli del regime di maggior tutela. State esponendo milioni di famiglie fragili di questo Paese a una vera e propria stangata a partire da gennaio 2024: altro che tutela del potere d'acquisto, altro che decreto bollette! *(Applausi)*. per proteggere le bollette degli italiani è totalmente assente, nonostante quello che chiedono l'opposizione e persino alcuni esponenti della maggioranza. quello che dovrebbe essere un decreto-legge per l'energia e per il potere d'acquisto è un decreto che parla di energia, ma anche di borse di studio, di caro materiali e di compagnie di assicurazione. È l'ennesimo decreto *omnibus*, ma soprattutto

Non ci sono interventi efficaci contro il caro energia, né una strategia per la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, che il Governo non è stato capace di mettere in campo nei primi dodici mesi di operato e di operato e che non vediamo nemmeno nella legge di bilancio, perché questi sono un Governo e una maggioranza che a parole sono vicini al popolo, ma quando si arriva alle scelte concrete stanno da un'altra parte. Neanche questo provvedimento sta dalla parte dei consumatori.

qualche collega in precedenza ha detto che era assente, ma mi pare che sia sempre stata presente e abbia svolto la sua relazione con estrema serietà e professionalità. Ho anche ascoltato alcune parole che mi hanno fatto riflettere, *in primis* quando una collega senatrice ha parlato delle sovrintendenze che bloccano le imprese che vogliono creare gli impianti. Io so solo una cosa: la sovrintendenza non fa altro che proteggere un bene costituzionalmente tutelato, quello del paesaggio. Se le sovraintendenze intervengono per bloccare delle imprese, significa che quelle imprese stanno violando il paesaggio, che è un bene protetto.

quando ho sentito parlare di merito. Per me merito significa partire tutti insieme e poi i più bravi vanno avanti. Qui invece ricordo che il merito per una forza politica era il reddito di cittadinanza, per cui Ricordo anche quell'episodio in cui l'allora Vice Presidente del Consiglio si affacciò sul balcone di Palazzo Chigi, mentre che loro avevano debellato la povertà con il merito, tramite il reddito di cittadinanza. Forse, prima di parlare è meglio riflettere su quello che si è fatto e che si è rappresentato in passato. Torno all'argomento di oggi. Il provvedimento all'attenzione odierna di quest'Assemblea si pone principalmente l'obiettivo di supportare le famiglie italiane con fasce di reddito basse per superare le problematiche legate alla quotidianità. Ad esempio, con attenzione verso le famiglie che non superano un ISEE di 15.000 euro, si concede una riduzione delle bollette di gas e luce. Possiamo quindi dire con forza che questo è l'ennesimo provvedimento che dimostra la vicinanza del Governo Meloni alle fasce deboli e alle famiglie. Questo Governo, non un altro, ha impegnato per il biennio 2022-2023 circa 30 miliardi di euro, che è più di quanto abbia fatto per la medesima finalità il resto degli Stati europei. Ricordo brevemente che già nella manovra finanziaria 2022 il Governo Meloni stanziava 21 miliardi di euro per contrastare il caro energia. Con questo decreto-legge si stanzia, per il supporto alle famiglie e alle fasce deboli, oltre 1 miliardo di euro, tra proroga delle misure per il caro energia, azzeramento degli oneri generali del gas e tanto altro. È tale l'attenzione di questo Governo, nel rispetto degli impegni assunti in campagna elettorale, che anche nella manovra finanziaria 2024 sono previste ulteriori misure a supporto delle famiglie più deboli. Tutto ciò nonostante le ristrettezze che ci impone il bilancio dello Stato, appesantito dagli sprechi cui abbiamo assistito nei Governi precedenti, uno su tutti il superbonus. Si tratta di una visione di Stato e di *welfare* che alle opposizioni non piace, ma ce ne faremo una ragione. Le opposizioni a questo Governo evidentemente preferiscono - scusatemi se lo ricordo, ma certe cose non devono e non possono essere dimenticate

che strumentalmente per le opposizioni non c'è un'emergenza carovita, non c'è necessità di aiutare le famiglie a pagare le bollette e non dobbiamo aiutare gli studenti con le borse di studio in un periodo in cui il potere d'acquisto delle famiglie è fortemente diminuito. Quando sento le opposizioni criticare questo decreto-legge, come se fosse l'origine di tutti i mali, mi sembra più chiaro perché gli italiani hanno scelto noi e non loro. Se la grande pecca di questo decreto, secondo le opposizioni, è che non prevede misure strutturali, permettetemi di puntualizzare una cosa: non è vero che questo Governo non sta costruendo le basi per affrontare la dipendenza energetica dell'Italia e per velocizzare la transizione energetica. energetica. Diciamo la verità agli italiani, diciamo che le misure strutturali che sta portando avanti il Governo Meloni, non certo con questo provvedimento che è un decreto d'urgenza, non è vero che non esistono, ma solamente non piacciono alla sinistra e non vi piacciono perché dopo dieci anni con il Governo di centrosinistra, illuminati dal MoVimento 5 Stelle, siamo al punto di partenza. Siete voi che non avete avuto il coraggio e la voglia di dare risposte serie al Paese. Le prove di una seria strategia sulla transizione energetica sono sotto gli occhi di tutti, basti pensare alle proposte di modifica formulate per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e al nuovo programma REPowerEU REPowerEU che è entrato in vigore lo scorso marzo e che prevede nel breve termine l'acquisto congiunto di gas, nuovi partenariati energetici con fornitori affidabili e una rapida realizzazione di progetti nell'ambito dell'energia rinnovabile, mentre nel medio periodo sono previsti l'integrazione nel PNRR, l'accelerazione della decarbonizzazione industriale e un nuovo quadro normativo per l'utilizzo dell'idrogeno. Il Governo è al lavoro per rendere l'Italia un *hub* europeo del gas e su questo punto dobbiamo dire la verità agli italiani: la 6a Commissione europea ritiene non bastevole l'energia prodotta da eolico e da fotovoltaico, tanto da aver deciso di includere gas e nucleare nell'elenco delle fonti rinnovabili, riconoscendole quindi come attività finanziabili. In questo dobbiamo riconoscere alla presidente Meloni l'intuizione della rotta da seguire con il suo piano Mattei, piano che porterà l'Italia a diventare il maggiore esportatore di gas naturale e di idrogeno verso Germania e Austria e acquisire centralità nel collegamento tra il Nord Africa e i Paesi dell'Europa centrale e settentrionale. Pertanto, quando si dice che il Governo non ha lungimiranza e non sta progettando interventi strutturali, si mente. Gli interventi strutturali non possono essere contemplati in un decreto d'urgenza, ma si inseriscono nel solco di altri provvedimenti come il REPowerEU, che quota circa 19 miliardi e che rappresenta una spesa corrente momentanea per esigenze momentanee, non dà una risposta strutturale sul fronte della sicurezza, dell'approvvigionamento di gas, della diversificazione degli approvvigionamenti, della incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e delle filiere industriali strategiche. Tra l'altro, queste cose le ha rimarcate in più occasioni, anche in quest'Aula, il ministro Fitto. La verità è che l'opposizione non accetta che per la prima volta l'Italia abbia un Governo serio nell'approccio delle strategie a lungo termine anche nel campo energetico. Approccio che è realistico e sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma economico e sociale. Infine, permettetemi una breve parentesi: quella che voi chiamate sanatoria o condono, noi la chiamiamo salvataggio di piccoli esercizi commerciali. Questa norma supera un disagio creato dalla prima applicazione di una nuova normativa sulla trasmissione dei corrispettivi in modalità elettronica. Parliamo di errori che non per forza sono compiuti con l'intento di evadere da parte di soggetti che esercitano attività di impresa. Ora, mi rendo conto che nella *forma mentis* di molti chiunque sia imprenditore, piccolo o grande, è evasore per eccellenza, ma non posso credere che anche tra i banchi dell'opposizione non sia chiaro che in sede di prima applicazione di quella norma ci sono stati confusione e problemi applicativi, dei veri e propri cortocircuiti che non sono certo addebitabili ai contribuenti. Sfido chiunque a dire pubblicamente che quelle errate trasmissioni siano tutte o in parte dolose. Consentire il ravvedimento operoso per per errori commessi in un periodo davvero limitato di tempo sulla trasmissione delle certificazioni in sede di prima applicazione non è sanatoria. Lo dobbiamo dire forte e chiaro, è lo Stato che da repressivo diventa lo Stato vicino ai contribuenti. Per questi motivi, non posso che annunciare senza tentennamenti il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.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

i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

dell'articolo unico del disegno di legge n. 937, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

è ieri, è tra un mese, è tutti i giorni. Si tratta di una questione che ha visto, negli ultimi fatti di cui le cronache ci fanno inevitabilmente partecipi, il brutale assassinio di Giulia Cecchettin ad opera del crudele compagno Filippo Turetta.

a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol, trascinandola lungo i vicoli e le strade della zona universitaria, fino ad arrivare sotto al portico di via dell'Unione e, dopo averla

mercoledì 15 novembre, e quindi solo qualche giorno fa, ha diffuso la notizia dell'abuso di una ragazzina di tredici anni mentre si trovava alla fermata dell'autobus.

quotidiano. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi e delle istituzioni affinché ci sia maggiore attenzione per prevenire, non per ricordare, non per parlarne solo il 25 novembre, perché ogni giorno è così e ogni giorno dobbiamo stare attenti perché fatti del genere non accadano. *(Applausi)*. ringrazio, senatore Amidei, credo che domani avremo occasione, oltre che di affrontare la discussione di un importante provvedimento, anche di mettere sul tavolo una serie di azioni e proposte proprio sul tema

sull'avvio di una procedura di infrazione sulla questione delle concessioni balneari. Questo significa due cose in particolare. La prima è una conferma che questo Esecutivo è inadeguato, incapace e pavido nell'affrontare il provvedimento e ha agito per difendere gli interessi di pochi a discapito degli interessi di tutti. Il bene di un Paese è stato piegato ai desideri di pochi.

di mettere in sicurezza chi ha un problema con la ludopatia, strizza l'occhio alle *lobby* dell'azzardo, aumentando le giocate del Superenalotto e facendo cassa su questo. Invece di tassare gli extraprofitti, come quelli delle banche, si va a aumentare l'IVA sui prodotti per l'infanzia e gli assorbenti per le donne; invece di aumentare la spesa sanitaria, si aumenta la spesa

Ciò significa gettare nel panico un intero settore strategico del nostro Paese, quello turistico, e tutto l'indotto che si crea intorno. Servivano certezze, soprattutto per i Comuni che dovevano andare alle procedure ad evidenza pubblica e dovevano avere certezza di come affrontare questo percorso.

Queste sono politiche fatte solo di parole. Dall'altra parte, si sta aiutando qualcuno, alcuni di quei concessionari particolarmente agiati che avranno la possibilità di avere le le coperture per poter intervenire sui bandi, partecipare e conquistare più spazio possibile; invece, i piccoli artigiani, i piccoli imprenditori che si volevano tutelare, saranno quelli più in difficoltà di tutti.